per tentata concussione (così recita la nota dell'agenzia), proprio stamattina, con una puntualità cui peraltro la magistratura ci aveva già abituato altre volte; vi sono già dei precedenti in tal senso. Mi dicono (almeno queste sono le notizie che circolano al momento) che il Ministro dovrebbe recarsi alla Camera questa mattina e rassegnare le proprie dimissioni. Al di là

aleggiare nell'aria: guarda caso, l'aria campana, dove di fumi ne abbiamo fin troppi in questi giorni. Devo ammettere che

fare il loro dovere al di sopra delle parti hanno sempre usato i potentissimi mezzi a disposizione della magistratura (soprattutto le procure) per fare politica anche nelle aule dei tribunali.

le dimissioni automatiche di un uomo politico, soprattutto di un Ministro, se viene colpito dalla magistratura perché, colleghi, questo vorrebbe dire che la classe politica, la classe parlamentare e governativa verrebbe scelta a quel punto automaticamente dalla magistratura. Questa

il capogruppo della Lega, il senatore Castelli, stamattina è stata arrestata per tentata corruzione

nelle persone dotate di un minimo senso della legalità e di rispetto delle istituzioni. Ieri abbiamo appreso dai giornali che la magistratura napoletana aveva disposto che fosse messo all'asta l'alloggio di un cittadino che non aveva pagato la TARSU, la tassa sui rifiuti. In pratica, questo cittadino napoletano, per non avere pagato la tassa sui rifiuti,

sanguinari esponenti delle più feroci famiglie camorriste sono regolarmente scarcerati per decorrenza dei termini.

A Napoli, la magistratura ritiene che le concessioni edilizie siano date non da chi governa la città, ma da rappresentanti dell'opposizione, che appunto vengono arrestati per le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Napoli.

nel corso del confronto sulla finanziaria.

Presidente, colleghi, certamente riesce difficile non sottolineare la straordinaria tempestività che si ripete nello scenario campano. infatti l'avviso di garanzia al presidente del Consiglio Berlusconi, in occasione del G8 di Napoli, quando si parlava della problematica della corruzione e della lotta alla criminalità. Guarda caso, quando il Ministro della giustizia deve riferire in Parlamento sullo stato dell'amministrazione della giustizia, improvvisamente arriva notizia di un provvedimento di arresti domiciliari nei confronti della moglie del Ministro, presidente del Consiglio regionale della Campania.

gettando certamente nello sconcerto tutti noi, perché sarebbe logico pensare che l'interessata sia la prima a dover sapere tutto ciò. Ed allora, delle due l'una: o è un *ballon d'essai* oppure è qualcosa di più grave e cioè il solito uso strumentale di una giustizia che arriva prima sui *media* e poi

c'è un problema di controllo complessivo di un sistema che sta impazzendo. Perché se è vero che il reato contestato alla signora Lonardo, alla presidente del Consiglio regionale della Campania, è di tentata - sottolineo "tentata" - concussione nei confronti di un soggetto, di un primario o di chi altri, ci troveremmo di fronte ad un reato la cui gravità

lieve nella considerazione ordinaria dei delitti che ne fa la magistratura se per tanti versi reati molto più gravi non vengono assistiti da provvedimenti cautelari altrettanto importanti.

un problema serio, che vede una magistratura inclinata verso un giustizialismo forte nei confronti della classe politica e meno forte - a parità di gravità di reati - nei confronti della criminalità organizzata,

Perché improvvisamente il procuratore Cordova, voluto dalla sinistra, viene cancellato dall'assemblearismo della procura di Napoli? Perché, oggi, viene colpito il Presidente del Consiglio regionale della Campania? C'è un attacco alla politica, o ad alcuna parte della politica, che appare fin troppo chiaro. C'è una tempestività che va valutata. Troppe volte, colleghi, ho visto politici arrestati non con provvedimento domiciliare ma tradotti in carcere e poi assolti con formula piena: nel frattempo il danno era stato fatto e le conseguenze si erano avverate, vale a dire l'attacco ad una determinata parte della politica. Penso che tutto questo debba finire. Ritengo che il Parlamento debba affermare la propria forza, la propria autonomia e la propria capacità di reagire senza toccare assolutamente, ripeto, princìpi costituzionali che sono alla base della nostra democrazia, ma certamente introducendo un sistema di vigilanza, di controlli che eviti queste forme di delegittimazione sempre e comunque, che alimentano - alla fine - un'antipolitica che è facile fare È facile, poi, fare di tutta un'erba un fascio e dire: "Quello è un politico, quindi è corrotto ad ogni costo". Perché sono questo tipo di azioni, questo genere di provvedimenti che non valutano le conseguenze

a conoscenza di un provvedimento della magistratura e, proprio per il rispetto della separazione dei poteri, dovremmo quantomeno attendere di sapere qualcosa di più. Credo che dovremmo in questo Paese riprendere la cultura della separazione dei poteri, nel senso che i poteri tra di loro dovrebbero riconoscersi vicendevolmente e legittimarsi, cosa che succede molto spesso in altri Paesi, succede molto spesso in altri Paesi, dove appunto la magistratura è anche criticata e attaccata, ma sui provvedimenti c'è poi un riconoscimento di questa separazione. Pensiamo alla Francia: Pensiamo alla Francia: non crediamo che i politici francesi siano immuni dalla critica o da provvedimenti giudiziari, né crediamo che la magistratura francese sia immune da critiche, anche violente,

e per quanto mi riguarda personalmente ad informarmi, dei pochi fatti che sono finora a nostra conoscenza. Sì, vorrei insistere su tale questione: i fatti sono pochi, ma salta ai nostri dell'opinione pubblica, che assiste a queste vicende, l'allarme determinato da un provvedimento restrittivo nei confronti della Presidente del Consiglio regionale della Campania. Si tratta di una decisione delicata e grave. Non conosciamo le indagini che sono alla base di tale decisione, né è nostro compito conoscerle, né censurare direttamente le iniziative di un'autorità giudiziaria. Tuttavia, è nostro dovere, fin dall'inizio io credo, di questa vicenda di cui vedremo gli sviluppi nelle prossime ore, ribadire un principio che è inderogabile: quanto più delicate sono le indagini giudiziarie in materia penale,

tanto più rigoroso deve essere, da parte delle autorità giudiziarie competenti, il rispetto delle regole: rispetto delle regole del diritto sostanziale, le quali chiedono una valutazione attenta attenta e seria delle condizioni di fatto, le quali possono corrispondere ad una figura astratta di reato prevista dal codice penale; allo stesso modo, rispetto delle regole processuali, fissate, tra l'altro (ma noi dobbiamo dire fondamentalmente) a garanzia del diritto alla difesa dei singoli cittadini che si trovino coinvolti in indagini o in procedimenti penali. Questi sono i princìpi che in questo momento dobbiamo richiamare. Aspettiamo gli sviluppi della vicenda, sapendo che esistono nel nostro Paese tutte le istituzioni, le garanzie e le regole relative alla divisione dei poteri, ma anche al controllo - necessario sull'attività delle autorità giudiziarie, entro e fuori l'ufficio e nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, tali da garantire la libertà dei cittadini e la tranquillità dell'opinione pubblica. L'allarme è, quindi, giustificato dai fatti di attualità, ma deve essere immediatamente compensato dalla freddezza con la quale richiamiamo tutti al rispetto delle regole. Questo il Senato può farlo, può farlo, in rappresentanza dei cittadini e del Paese, e per le funzioni di controllo proprie di una assemblea parlamentare. È dunque con serenità che dobbiamo affrontare questa come altre vicende, senza decampare dai princìpi fondamentali del nostro agire e da quelli che devono ispirare un'istituzione come il Senato, nell'ambito del rispetto rigoroso delle regole della Repubblica.

La vicenda giudiziaria dovrà svolgersi ragionevolmente nel più breve tempo possibile, ma non ha alcuna connessione con la vicenda dei rifiuti in Campania. Non sottovalutiamo il fatto che si tratta della moglie del Ministro della giustizia. Non riteniamo vi sia alcuna ragione per la quale il Ministro debba dimettersi. Riteniamo che l'autonomia della magistratura vada in questo caso rispettata. Capiamo che la decisione della magistratura di oggi può influire sulla vicenda politica in modo notevole. Non riteniamo che possa essere stato estranea all'orientamento del giudice questa valutazione politica, ma intendiamo ribadire in questo momento la convinzione dell'UDC

di fronte agli studenti americani e subire anche le critiche da parte degli stessi. Le istituzioni italiane non sono riuscite a garantire che ciò accadesse in un'università

al giudice De Magistris che subì quel provvedimento disciplinare. Ora, correlare sarebbe ingiusto e probabilmente anche sbagliato, ma questo fatto

viene colpito, per un sospetto di tentata concussione, il Presidente del Consiglio regionale che viceversa, se dovesse cadere per le sue dimissioni, non trascinerebbe con sé né il Consiglio regionale né il Comune di Napoli.

a violare il principio di separazione. I fatti a nostra conoscenza non sono sufficienti per esprimere alcun giudizio e alcuna valutazione. Rispettare l'autonomia della politica vuol dire anche evitare di aprire improvvisati e frettolosi dibattiti e, per quanto riguarda gli esponenti politici, evitare di prendere frettolose decisioni sull'onda di provvedimenti di questo tipo.

Signor Presidente, le notizie delle agenzie di stampa sono così scarse che non consentono a nessuno di noi di esprimere giudizi. Per abitudine, tutte le volte che interviene la magistratura, io non commento. Si tratta, però, di una vicenda estremamente grave perché va a colpire la famiglia del Ministro della giustizia e nessuno di noi può sottovalutare tale aspetto.

riportando le agenzie, quando si scrive "tentata corruzione" o "concussione" e con una tentata concussione automaticamente si procede all'arresto,

per capire come uscire da questa situazione di declino sconcertante, che ci rende ridicoli di fronte al mondo intero.

aspettiamo che la magistratura faccia il suo corso e vogliamo esprimere solidarietà umana al ministro Mastella, aspettando che egli stesso faccia, secondo coscienza, le valutazioni che riterrà più opportune.

che, letta dall'esterno (come succede a tutti noi), è, obiettivamente, sconcertante. Sono d'accordo con i colleghi che reclamano quel principio d'indipendenza e di autonomia, che è fondamentale. Io, però, vorrei vivere in un Paese dove l'autonomia dei magistrati fosse un valore assicurato così come fosse assicurato un altro principio, quello dell'autonomia della politica dalle ingerenze dei magistrati. Dico ciò perché, in base alle poche notizie che ci giungono, rispetto a una contestazione di questo tipo forse qualche disvalore è stato messo in campo. La sensazione di sgomento viene chiaramente aumentata dal fatto che, molto spesso, in Commissione giustizia

che molto spesso, per cause che comunque fanno riferimento alla sfera giudiziaria, vengono calpestati. Signor Presidente, vorrei immaginare di vivere in un Paese nel quale la dignità di ognuno viene garantita accanto all'indipendenza della magistratura. Ma - lo devo proprio dire - in un giudizio di valore preferisco che la dignità di ognuno prevalga su tutti gli altri princìpi.

i relativi emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.101 e 7.0.100, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 1 dell'articolo 4, secondo periodo, siano soppresse le parole: "di 200.000 euro per l'anno 2007 e" e che il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. All'onere recato dal comma 1, pari a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008‑2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute". Esprime altresì parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.102, 5.5 e 1.0.100, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e della proposta 5.104, sulla quale il parere è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione dopo le parole: "selezione costituiti"

suggerisce, se non vi sono motivi ostativi, di procedere all'esame dell'articolo 2, accantonando temporaneamente l'articolo 1. Chiedo

il testo oggi non venisse modificato, si cambia in corso d'opera una situazione giuridica già prestabilita, tanto che il mio emendamento è analogo a quello del senatore Adragna e di altri componenti, sia della maggioranza sia dell'opposizione: è un discorso di carattere generale. Mi auguro che la relatrice ed il relatore siano favorevole a questo emendamento.

per tutte le istituzioni di alta formazione artistico-musicale. Ma lo stesso decreto, con una norma transitoria all'articolo 16, prevede che i direttori dell'Accademia di arte drammatica e dell'Accademia di danza in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono le funzioni fino alla cessazione del rapporto per effetto del verificarsi di cause previste dalla normativa vigente. In questo modo è stato riconosciuto ai due direttori un diritto acquisito, che adesso si vorrebbe conculcare senza alcuna motivazione. È opportuno ricordare che questa norma, oltre a ledere il pacifico principio dell'affidamento contrattuale, ricalca norme recenti, la più importante delle quali è l'articolo 3, comma 7, della legge n. 145 del 2002, quella sul cosiddetto *spoils system*, che un'importante sentenza della Corte costituzionale, la n. 103 del 2007, ha definitivamente bocciato nella parte in cui prevede la cessazione immotivata ed automatica di incarichi dirigenziali. Infatti, la Corte ha stabilito che la cessazione delle funzioni dirigenziali può essere disposta dalla legge solo in presenza di accertata responsabilità del funzionario dirigenziale, in presenza di determinati presupposti, e all'esito di un procedimento di garanzia. Solo un legame tra cessazione della carica e valutazioni oggettive dell'attività dirigenziale può legittimare il legislatore a rimuovere un dirigente dall'incarico espletato. Alla luce delle suddette considerazioni, il comma 2 dell'articolo 5, così come formulato, è a mio avviso incostituzionale, contrasta con le più recenti decisioni della Corte e darebbe senza dubbio luogo a pesanti oneri risarcitori dello Stato, così come sta avvenendo nel contenzioso originato dalla legge n. 145 del 2002.

Essa dunque non ha quei caratteri di astrattezza e generalità che si richiedono alle leggi di un ordinamento democratico e garantista, anzi ha il carattere di una legge provvedimento, cioè di una norma che, che, nella sostanza, è un provvedimento amministrativo di carattere repressivo. Quindi, a maggior ragione, si tratta di una norma che dovrebbe essere corredata da un'adeguata motivazione e contro la quale i diretti interessati non dispongono delle tutele giurisdizionali ordinarie che la nostra Costituzione, all'articolo 24, riconosce a chi si ritenga leso in un proprio diritto o in un proprio interesse. *(Congratulazioni)*.

parere del Governo è conforme a quello del relatore. Mi permetta, Presidente, di aggiungere una parola riguardo all'emendamento 5.2, per motivare il nostro invito al ritiro. Comprendiamo le ragioni di contrarietà al problema dell'intermediazione sul mercato del lavoro. caso si tratta, però, di risolvere un problema tecnico estremamente limitato. La normativa vigente presenta infatti un'anomalia: permette di svolgere attività di intermediazione alle università, ma non ai loro consorzi. una norma che non aiuta la semplificazione dell'azione amministrativa e la presenza consortile degli atenei in questo campo. Quindi, la contrarietà e l'invito al ritiro vogliono sollecitare la senatrice Capelli

a trovare la copertura economica necessaria per realizzare l'equiparazione del trattamento tra i docenti universitari che svolgono le stesse funzioni del personale ospedaliero e che oggi sono ingiustamente discriminati.

di un problema annoso, che si trascina da troppo tempo e che determina un'ingiustificata discriminazione a danno dell'università. Chiedo per l'ennesima volta a questo Governo di non penalizzare l'università italiana e la ricerca, come purtroppo in questa legislatura ha costantemente fatto; si prenda carico una volta per tutte del problema università che in questo Paese, purtroppo, dall'attuale Governo è del tutto disatteso. *(Applausi dai Gruppi AN e ci dispiace molto che non sia possibile in questo momento approfondire il senso ultimo dei due emendamenti che abbiamo presentato, che attiene al problema della legge n. 30 del 2003 e del lavoro precario, ed in modo particolare alla precarizzazione del lavoro intellettuale di chi esce dalle università.

grandi battaglie in Parlamento. Dispiace, quindi, che non sia possibile approfondire il dibattito e che il parere del Governo si sostanzi in un invito al ritiro. Tenendo conto, però,

laddove poneva un presidio all'esercizio della funzione di collocamento da parte della singola università. La funzione di collocamento, nell'intenzione del legislatore, dovrebbe essere funzionale a dar luogo ad un canale di dialogo interattivo con il mercato del lavoro e l'economia del territorio circostante, non soltanto, quindi, in funzione dell'erogazione di un servizio d'incontro tra la domanda e l'offerta (servizio rivolto agli studenti di quella università). La delega ad un consorzio diventa altra cosa. Diventa un modo con il quale l'università rinuncia a svolgere quella funzione delegandola ad una soggetto terzo e lontano, in certa misura estraneo, al rapporto con il territorio circostante, con l'economia, con il mercato del lavoro nel quale l'università è inserita. Questa è la ragione di quel divieto. Altri soggetti possono farsi autorizzare secondo le procedure che la legge prevede perché la legge Biagi non dispone la liberalizzazione della funzione del collocamento ma, nel momento in cui la rende plurale, la sottopone ad un rigoroso regime autorizzatorio con richiesta di capitale sociale e requisiti per gli amministratori. Quindi i soggetti che in passato si sono organizzati come consorzi universitari possono ancora farlo, ma non sulla base di una delega dell'università, dando vita a società debitamente capitalizzate e i cui amministratori devono possedere i requisiti che la legge prevede. Per questa ragione chiediamo il ripristino del testo originario della legge Biagi.

Senz'altro riconosciamo l'interesse specifico e la capacità delle università di svolgere quelle attività, ma se si ammette questo il consorzio universitario,

molto strano e incongruente che non si permetta a consorzi di università di esercitare la funzione di intermediazione.

circostante le Marche. Nella fattispecie, l'unico consorzio esistente e funzionante in Italia è quello di AlmaLaurea che copre 50 università, che ha nella propria banca dati quasi un milione di *curriculum* di laureati italiani, che ha diffuso presso le imprese mezzo milione di questi *curriculum*, che sta estendendo la propria attività ad università straniere e che quindi è in contatto con un mercato del lavoro

che è largamente condiviso il tentativo di porre rimedio ad una paradossale ingiustizia determinatasi nei confronti di circa 300 laureati in medicina e chirurgia

l'esame di abilitazione all'esercizio della professione per questi laureati è stato fissato 15 giorni dopo la data di scadenza del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione. Contrariamente a quanto avvenuto nel passato, non è stato consentito a questi laureati di accedere al concorso, riservandosi di produrre successivamente l'ottenimento della prescritta abilitazione. Anzi, il TAR ha riconosciuto questo diritto e li ha ammessi con riserva. Questi laureati hanno sostenuto il concorso, sono risultati vincitori, ma nel momento in cui dovevano avviarsi all'attività didattica che iniziava a settembre (dunque, avendo già conseguito la prescritta abilitazione) il Consiglio di Stato ha ritenuto invece di non condividere la decisione del TAR e ne ha quindi decretato l'esclusione. La situazione è ora assurda, perché i vincitori del concorso non possono partecipare, mentre gli idonei, al loro posto, si sono visti avere la possibilità di accedere. Ma la situazione è ancor più paradossale, perché moltissimi posti di quel bando sono rimasti scoperti per assenza di idonei e altri sono rimasti scoperti pure in presenza di idonei, perché non ve ne erano in misura sufficiente a coprire tutti i posti. Quest'anno, signor (situazione che rende ancora più opportuno l'emendamento), il Ministero ha giustamente anticipato l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di medico prima della scadenza del bando di accesso alle scuole di specializzazione, ha consentito di poter partecipare anche con riserva potendo presentare successivamente il titolo e addirittura la legge finanziaria di quest'anno consente perfino ai non laureati di partecipare, riservandosi di produrre la documentazione alla alla data successiva alla scadenza del bando di accesso alle scuole di specializzazione. Solo a questi 300 studenti laureati in medicina e chirurgia verrebbe dunque impedito l'accesso alle scuole di specializzazione. Con l'emendamento in esame si pone rimedio a questa evidente ingiustizia e chiedo al relatore, al Governo e ai colleghi senatori presenti in quest'Aula di acconsentire, con il loro parere e il loro voto, affinché l'emendamento venga approvato.

infatti era previsto il concorso per la specializzazione a gennaio e l'esame di abilitazione a febbraio, il che significava sostanzialmente che i ragazzi che si erano laureati a luglio dovevano aspettare un anno e mezzo prima di accedere alla specialità. Ciò era un'autentica porcheria; mi scusi il termine, signor Presidente, ma credo sia

alla fine si è arrivati ad una conclusione che consente per quest'anno a quei ragazzi di non perdere la possibilità di accedere alle scuole di specializzazione. A questo punto si viene però a creare una palese discriminazione rispetto a coloro che l'anno scorso hanno subito un analogo trattamento,

Mi pare assolutamente evidente che, secondo un principio di equità, si debba votare questo emendamento; soprattutto, teniamo sempre presente che abbiamo a che fare con la carriera, con la vita, con le prospettive lavorative di giovani bravi, che non possono essere penalizzati. Se poi, per avere il consenso del senatore Tomassini, si vuole eliminare la parola «anche», personalmente sono d'accordo. Proporrei allora una riformulazione, chiedendo ai colleghi che hanno presentato l'emendamento di sopprimere

perché sappiamo come finiscono: cominciano le catene dei vari avvocati che telefonano a tutti i medici specializzati e prende l'avvio un processo che sicuramente non va a vantaggio né degli specializzandi né dei futuri pazienti.

Presidente, ritengo di eliminarla proprio per equità nei confronti degli accessi alle scuole di specializzazione. Non vi è dubbio che, detto così ("in soprannumero"), la spesa aumenterà.

il Governo è comunque favorevole.

non è vero che si creerebbero disparità di trattamento); inoltre, talvolta nelle scuole di specializzazione rimangono posti vacanti, per cui non è necessario che tutti siano in soprannumero perché alcuni possono rientrare anche nei posti che rimangono vacanti.

Presidente, apprendiamo adesso che il ministro della giustizia Mastella si è appena dimesso. La motivazione è quella di cui abbiamo discusso questa mattina, cioè i gravi fatti che hanno coinvolto la moglie, ma è indubitabile che in questo momento ci troviamo di fronte ad una grave emergenza e ad una grave crisi istituzionale. Le parole del ministro Mastella, almeno da quanto apprendiamo dalle agenzie, le seguenti: «Mi trovo in una situazione di paura». È una parola che non abbiamo mai sentito pronunciare da un Ministro fino ad oggi

Non ho le stesse motivazioni che ha esposto la senatrice Alberti Casellati. Il tema della paura è un problema che riguarda la persona che si sente colpita da questo sentimento, da questo senso di angoscia. che l'amministrazione della giustizia deve essere guidata da chi è al di sopra di ogni sospetto e, a maggior ragione, deve esserlo la moglie di Cesare. Credo che le dimissioni del Ministro della giustizia siano un fatto grave nella vita di un Paese. Stiamo parlano

Credo che sia il Presidente del Consiglio a dover riferire all'Aula se intende andare avanti con l'azione di Governo. Tutte le discussioni fatte fino adesso,

*(AN)*. Signor Presidente, credo che non debba fare grandi riflessioni per denunciare

Peraltro, non è la prima volta che il ministro Mastella denuncia problemi relativi alla propria persona e, quindi, alla propria incolumità.

di quest'Aula, o comunque del Parlamento, ma rappresentano il clima importante in cui la politica oggi deve vivere e, oserei dire, sopravvivere. Pertanto, presidente Calderoli, va da sé che la richiesta prioritaria non è quella di concludere un provvedimento (che, tra l'altro, non rappresenta neanche il campo di Marte per quanto riguarda i soggetti

che, da oggi e nei prossimi giorni, si dovranno fare in riferimento al Governo della nostra Nazione, nei confronti della quale abbiamo ampia dedizione ed impegno.

credo che se le parole pronunciate dal ministro Mastella sono quelle riferite dalla collega Alberti Casellati, se cioè il Ministro ha paura, siamo in presenza di una questione di estrema gravità istituzionale. Non si tratterebbe della paura per un attentato o per un incidente stradale, ma sembrerebbe di capire che il Ministro della giustizia - che non è persona irresponsabile e al quale confermiamo la richiesta di non insistere sulle dimissioni, anche se la questione è molto delicata

Signor Presidente, sono già intervenuto sull'argomento e adesso che - confesso - mi sono assentato dall'Aula per ascoltare di persona il discorso del ministro Mastella,

peraltro mi onoro di essere amico, che sono dei gran signori, oltre che signori del diritto, della libertà e delle garanzie. Ve ne sono, però, altri che di fatto fanno politica e usano il loro potere

comunque, rimettiamo al Presidente della Repubblica le scelte per questa circostanza. Come possiamo continuare a parlare di emendamenti di fronte a questo stato di cose nel Paese? Vi

Presidente, le dimissioni del ministro Mastella rappresentano un fatto molto serio noi lo valutiamo come fatto di straordinaria responsabilità politico-istituzionale, oltre che di tutela, ovviamente, dell'onorabilità propria e della propria famiglia. Manifestiamo piena solidarietà al ministro Mastella, ricordando che le dimissioni non erano atto né dovuto, né richiesto da nessuno.